Ricordo che, ai sensi della Disposizione transitoria del Regolamento del Senato per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XVI Legislatura, il Gruppo Italia dei Valori ha avanzato la richiesta dì procedere all'elezione di un senatore Segretario. Su tale richiesta si è espresso in senso favorevole il Consiglio di Presidenza. Per effetto dell'accoglimento di detta richiesta, risulterebbe alterato a sfavore dei componenti dei Gruppi di maggioranza il rapporto numerico, in seno al Consiglio dì Presidenza, tra questi e i componenti dei Gruppi di opposizione; pertanto si procede, ai sensi del comma 2 della citata Disposizione transitoria, alla contemporanea elezione di un ulteriore senatore Segretario. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2*-ter*, del Regolamento, ciascun senatore scriverà sulla propria scheda un solo nome. Risulteranno eletti coloro che, essendo iscritti al Gruppo richiedente e a uno dei Gruppi di maggioranza, otterranno il maggior numero di voti, limitatamente a uno per ciascuno dei predetti Gruppi. Il numero totale dei senatori eletti non potrà comunque essere superiore a due. A parità di voti sarà eletto il più anziano di età. I senatori, chiamati in ordine alfabetico, passeranno sotto il banco della Presidenza e deporranno la scheda nell'urna predisposta.

Alicata, Allegrini, Amati, Amato,

Asciutti, Astore, Augello,

Bastico, Battaglia, Belisario, Benedetti Valentini,

Bosone, Bricolo, Bruno,

Caforio, Cagnin, Calabrò,

Caligiuri, Camber, Cantoni, Carlino, Carloni, Carofiglio, Carrara,

De Angelis, De Eccher, De Feo, De Gregorio, De Lillo, De Luca, De Sena,

Del Vecchio, Della Monica, Della Seta,

Ferrara, Filippi Alberto, Filippi Marco, Finocchiaro, Fioroni,

Fleres, Fluttero, Follini,

Franco Vittoria Galioto, Gallo,

Gentile, Germontani, Ghedini,

Giai, Giambrone, Giaretta, Giordano, Giovanardi, Giuliano, Gramazio, Granaiola, Grillo

Latronico, Lauro, Leddi,

Marinaro, Marini, Marino

Mazzuconi, Menardi, Mercatali, Messina, Micheloni, Milana,

Palma, Palmizio, Papania, Paravia, Pardi, Passoni, Pastore, Pedica, Pegorer, Pera,

Peterlini, Piccioni, Piccone,

Piscitelli, Pistorio, Pittoni, Poli

Rizzi, Rizzotti, Roilo,

Rusconi, Russo, Rutelli

Serafini Giancarlo, Serra, Sibilia, Sircana, Soliani, Soliani, Spadoni Urbani, Speziali,

Tomaselli, Tomassini, Tonini, Torri,

Grazie Vaccari, Valditara, Valentino, Vallardi, Valli,

Vimercati, Vita, Vitali, Vizzini Zanda,

nuova finestra"). Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta odierna, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide: per la Regione Lombardia, Marilena Adamo, Irene Aderenti, Emanuela Baio, Fiorenza Bassoli, Lorenzo Bodega, Daniele Bosone, Alessio Butti, Roberto Calderoli, Giacomo Caliendo, Gianpiero Carlo Cantoni, Giuliana Carlino, Valerio Carrara, Antonino Caruso, Mauro Ceruti, Ombretta Colli, Romano Comincioli, Riccardo Conti, Gerardo D'Ambrosio, Marcello Dell'Utri, Gianpiero De Toni, Cinzia Maria Fontana, Maria Alessandra Gallone, Guido Galperti, Pierfrancesco Emilio Romano Gamba, Massimo Garavaglia, Pietro Ichino, Giuseppe Leoni, Alfredo Mantica, Mario Mantovani, Rosa Angela Mauro, Sandro Mazzatorta, Alfredo Messina, Cesarino Monti, Roberto Mura, Guido Possa, Fabio Rizzi, Giorgio Roilo, Paolo Rossi, Antonio Rusconi, Salvatore Sciascia, Giancarlo Serafini, Antonio Tomassini, Tiziano Treu, Giuseppe Valditara, Armando Valli, Umberto Veronesi e Luigi Vimercati. Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Grazie

Presidente, vorrei solo informare, o ricordare, all'Assemblea che il 12 novembre scorso il Gruppo di alto livello istituito dall'Unione europea per la riduzione degli oneri amministrativi ha emanato un documento, il *Decalogue for Smart Regulation* (Decalogo per la buona legislazione) che invita i legislatori nazionali ad attenersi ad alcuni principi cardine di chiarezza, semplicità, concisione, sobrietà, comprensibilità e proporzionalità del numero e del volume delle norme rispetto alla materia trattata. Ora, l'emendamento che stiamo per votare riguarda una materia sulla quale solo tre settimane fa questo Senato ha

il collegato alla finanziaria n. 1167 entrerà in vigore a ruota entro gennaio (come la maggioranza preannuncia), la norma emanata oggi verrà abrogata implicitamente e sostituita da una norma che regolerà la stessa materia in modo diverso. Quando, proprio su questo punto, nel corso della discussione sul collegato alla finanziaria, abbiamo contestato questo modo disordinato di legiferare, il collega Castro ci ha risposto che questa va considerata come "stratificazione virtuosa".

nel fatto che il Governo tenda a rendere inemendabili le proprie proposte di legge da parte del Parlamento, questo dovrebbe consistere, quantomeno, nel fatto che le leggi siano semplici, coerenti, magari sbagliate, ma scritte bene e rispettose dei principi di organicità, chiarezza e comprensibilità. Qui, invece, se il Presidente mi consente di usare un'espressione poco aulica, «cornuti e mazziati», perché siamo espropriati della possibilità di emendare, ma ne siamo espropriati in funzione di leggi che sono caotica disorganicità gettano sostanzialmente sabbia negli ingranaggi della società civile e del tessuto produttivo. Questo è il risultato di una legislazione così disordinata e disorganica.

Spesso e volentieri tali provvedimenti sono stati oggetto di revoca, come è accaduto il 6 giugno scorso, quando il Presidente del Consiglio ha revocato l'ordinanza di sospensione del pagamento delle entrate. Il TAR

lo stesso meccanismo utilizzato per Umbria e Marche, cosa che oggi non avviene. La differenza è abissale: 12 anni di sospensione per Umbria e Marche, nove mesi per l'Abruzzo; 40 per cento di pagamento richiesto per Umbria e Marche, 100 per cento per l'Abruzzo;

Signor Presidente, dei 9 miliardi di euro che la manovra ha visto aggiunti con il passaggio alla Camera in seconda lettura nessuna risorsa è stata destinata al finanziamento di infrastrutture, nonostante la natura delle risorse reperite sia stata chiaramente *una tantum* e fosse chiaramente da finalizzare ad investimenti. Ebbene, nessuna risorsa è stata allo scopo destinata, ad eccetto della ricapitalizzazione della Società Ponte sullo Stretto, che rappresenta proprio quanto di più inopportuno e di più insensato si potesse fare. Di fronte all'immagine, anche plastica, di un Paese che letteralmente frana - dalle frane sistematiche e strutturali che si registrano sui cantieri della Salerno-Reggio Calabria a quelle più recenti dì Giampilieri a Messina - continuate scelleratamente ad insistere ostinatamente, come per la vicenda Alitalia, nel perseguire le promesse di una campagna elettorale che fu buona per una politica degli annunci fatta di *spot* efficaci mediaticamente, ma assolutamente avulsa dal contesto reale delle cose. Realizzare il ponte sullo Stretto, anche con una soluzione architettonica meno ardita di quella pensata per un ponte lungo oltre 3 chilometri a campata unica, su cui non poche sono le perplessità manifestate, significa allo stato reale e attuale delle cose collegare due deserti dal punto di vista infrastrutturale. Non abbiamo bisogno di opere faraoniche, né di cattedrali nel deserto. Con questo emendamento intendiamo richiamarvi alle vostre responsabilità e opportunamente vi offriamo la possibilità, in questa fase, tanto delicata per il Paese e in particolare per il Meridione - che non vedrà certo risolti i suoi problemi con l'istituzione della Banca per il Sud - di fare davvero qualcosa di utile per l'immediato e per il futuro più prossimo. Chissà che forse, così facendo, non si possa fare bene anche per la prospettiva realizzativa di quel ponte, forse, in quel caso, davvero materializzazione reale di tante legittime aspettative e aspirazioni. Non si edifica una casa dal tetto, ma dalle fondamenta! Questo è quello che noi sommessamente vi proponiamo con questo emendamento, destinando le risorse stanziate per la ricapitalizzazione della Società Ponte sullo Stretto alla realizzazione delle opere di completamento relative ai corridoi 1 e 8, che peraltro ci hanno già visto comunemente concordi nel riconoscerne la priorità in ripetuti ordini del giorno approvati dal Senato. Occorre prima del ponte - non al posto o in sostituzione di questo: soltanto prima, come vi chiediamo con questo emendamento - la realizzazione delle opere di adeguamento stradale e ferroviario nelle Regioni Sicilia e Calabria. È esclusivamente nell'interesse generale del Paese che vi chiediamo di approvare questo emendamento e di cambiarne la valutazione nel parere.

Signor Presidente, questa prossime festività natalizie saranno ricordate, oltre che per le nevicate eccezionali, anche per le intemperie sociali, che definirei gli effetti collaterali di una crisi internazionale che si dice in via di superamento. Mi riferisco alle tribolazioni di chi ha perso e di chi perde il lavoro, di chi lo cerca e non lo trova. non lo trova. Penso al nostro Mezzogiorno e alle tante risorse che sarebbero dovute per legge e che invece, con le ultime leggi finanziarie, sono state sottratte. Penso all'Italia, che celebra l'anniversario dei 150 anni di unità ed è sempre più divisa a metà. infine alla mia Regione, alla Campania, dove solo negli ultimi tre mesi sono andati perduti 20.000 posti di lavoro. Signor Presidente, signor Vice Ministro, di questi nostri lavori parlamentari e di questa legge finanziaria, invece, non si ricorderà molto, a parte i tanti «vorremmo, ma non possiamo», «sarebbe bello», «ci piacerebbe» che abbiamo sentito dal Governo. Allora, si potrebbe forse fare qualcosa che invece abbia un chiaro segno di sensibilità sociale di fronte a tanto disagio. Con l'emendamento 2.91 noi vogliamo reintrodurre il credito d'imposta, limitatamente alle Regioni del Mezzogiorno, per le imprese che assumono a tempo indeterminato e per un valore di 333 euro al mese per al mese per i prossimi tre anni. Inoltre, vorremmo introdurre un'ulteriore agevolazione per quelle imprese che incrementano l'assunzione di lavoratrici donne fino a 416 euro mensili per i prossimi tre anni. Signor Presidente, signor Vice Ministro, si potrebbe davvero fare e, dunque, per noi si deve fare. Sarebbe una decisione giusta; sarebbe una decisione benedetta.

«La cooperazione non funziona, e quindi non solo non lasciamo questi soldi, ma il prossimo anno togliamo anche quelli»; buonista: «La cooperazione ha funzionato troppo bene e quindi dobbiamo occuparci delle *leadership*, magari di Gheddafi, invece che occuparci dei denari»; tipo: «Il mondo è cambiato: siccome abbiamo bisogno di soldi, consideriamo i soldi che abbiamo tolto come un anticipo su quelli che chiederemo nei prossimi anni ai Paesi in via di sviluppo». Ecco tre altre ragioni che magari il nostro Vice Ministro potrà utilizzare per spiegare come mai siamo al punto più basso degli ultimi dieci anni.

Signor Presidente, vorrei approfittare della presenza del ministro Bondi, che non so se sia Ministro, si tratta di un emendamento, peraltro reiterato, che tende ad alleviare i tagli al Fondo unico per lo spettacolo. Lei sa che in questo momento c'è un'agitazione in corso, uno sciopero indetto a fronte di un taglio ormai inesorabile che sta portando alla chiusura decine e decine di compagnie.

il voto al Senato non trova giustificazione nel tanto sbandierato ostruzionismo delle opposizioni, visto che di ostruzionismo le opposizioni non ne hanno fatto e che queste hanno concentrato le loro proposte politiche solo ed esclusivamente su pochi emendamenti, compatibili e coerenti con le esigenze della finanza pubblica. Quindi, neanche quest'arma spuntata dell'ostruzionismo vi è giovata ad ammannire a questo Parlamento e a questo Paese una finanziaria che, per renderle onore, bisognerebbe chiamare inutile. Gran parte degli emendamenti che il nostro Gruppo parlamentare ha presentato, in prima lettura al Senato e in Commissione alla Camera, sono stati ritirati, infatti, per tenerne in piedi solo poche decine, i più significativi, che vertevano su questioni fondamentali, secondo noi, per il bene del Paese, a partire da una nuova politica fiscale per la famiglia. Di questi emendamenti non avevamo la presunzione di ottenere l'approvazione, ancorché auspicabile, considerata la loro ragionevolezza nel merito e l'urgenza del loro contenuto per garantire coesione sociale e ripresa economica, ci saremmo augurati che su di essi venisse avviato un confronto serio articolato. Questo confronto non c'è stato e ciò, dal nostro punto di vista, rappresenta motivo di particolare rammarico, unitamente alla circostanza che non è stato possibile esaminare a fondo il provvedimento in seconda lettura alla Camera in ragione del voto di fiducia. Perché questo modo di approvare la finanziaria? Forse perché fiducia. Perché questo modo di approvare la finanziaria? Forse perché

noi riteniamo che questo sia frutto dei contrasti che esistono, che sono evidenti sono emersi, anche con la presentazione di emendamenti in prima lettura al Senato e poi alla Camera, all'interno della maggioranza. Ci troviamo di fronte ad una maggioranza divisa in un dibattito un po' stucchevole, superficiale e artificioso fra i presunti tutori

non si riesce a capire quale sia e quale possano essere la vera politica economica di questo Governo e l'utilità di strutture anche interne alla Presidenza del Consiglio che si occupano di presunte politiche per la famiglia, inesistenti e inconcludenti. La verità è che noi ci troviamo di fronte ad un Governo che al suo interno ha profonde divisioni sul piano della politica economica e che ha scelto la strada del tirare a campare e di non incidere sull'andamento strutturale dei conti pubblici per evitare di rendersi impopolari, che, comunque, fa parte della responsabilità di chi ha la guida del Paese. Rispetto a questo, riteniamo che

di cui ha sempre dichiarato l'urgenza, a cominciare da quelle delle pensioni e del *welfare* in generale, per siglare un nuovo patto generazionale, della pubblica amministrazione (è di oggi la notizia di un

Grazie palesa come il Governo non abbia una strategia economica per il Paese. Essa si annunciava *light*, mentre incide e pesa per 9 miliardi di euro sui cittadini italiani.

che poi coprite con la finanziaria successiva perché altrimenti i buchi di bilancio renderebbero comunque paralizzante ogni attività del Governo con riferimento al bilancio dello Stato. Questa finanziaria è inefficace e insufficiente in quanto, tra l'altro, trascura tre questioni fondamentali

non avrà alcun effetto concreto per il Sud d'Italia, se non quello di fare l'ennesimo annuncio in danno della sottrazione permanente di risorse in favore del Mezzogiorno che voi state facendo da un anno e mezzo, a cominciare dai cosiddetti fondi FAS. Dove sono le misure annunciate dal Governo a sostegno di famiglie, pensionati e imprese? Dove è finito il piano per il Mezzogiorno, di cui resta solo un'ipotetica Banca del Sud e l'uso dei FAS per ripianare il debito sanitario? Dove è il piano per l'occupazione e la riforma degli ammortizzatori sociali? Dove sono le risorse per garantire effettiva sicurezza ai cittadini, che servirebbero molto più delle campagne di intolleranza di cui siete diventati campioni? Signor Presidente, siamo davvero preoccupati per il domani del nostro Paese; siamo preoccupati di dover lasciare ai nostri figli un Paese peggiore rispetto a quello che abbiamo.

Signor Presidente, anche quest'anno con la sessione di bilancio si chiude una dannosa e insostenibile commedia. Il copione, signor Vice Ministro, è sempre lo stesso: pochi articoli iniziali, accompagnati da fiumi di parole in cui vengono date lezioni magistrali di cosa sia un processo di modernizzazione di bilancio; poi, all'improvviso, spunta un maxiemendamento in cui si infila di tutto e di più, e poi, per paura del confronto, si paralizza il dibattito parlamentare con questioni di fiducia e bocciando gli emendamenti. Questa volta il ministro Tremonti ha superato se stesso, nemmeno Quintino Sella avrebbe saputo fare di meglio: in poco più di dieci giorni si è passati da niente a quasi 9 miliardi di risorse per misure confuse, contraddittorie, inadeguate e a tratti vergognose. nella sua ripetitività, ha finalmente fatto capire una cosa agli italiani: la vera questione, il vero limite non sono i vincoli di bilancio o il reperimento delle risorse, ma la debolezza politica di una maggioranza divisa al suo interno, in modo comico o tragicomico, tra chi sa già del fallimento del ministro Tremonti ma non può dirlo, e chi lo sa e lo dice, lo traduce in emendamenti, in disagi, in prese di distanza. Il problema è tutto qui. Nonostante i nostri sforzi e le nostre proposte emendative, non riusciamo a trovare una sola ragione perché questa finanziaria possa essere approvata. Da parte del Governo non si può continuare ad utilizzare solo gli strumenti degli indicatori di analisi economica; non si può far vivere gli italiani di percentuali sul PIL, di quadri tendenziali, di saldi netti da finanziare, perdendo di vista la concretezza dei problemi e il bisogno di un rapporto diretto e reale con la vita quotidiana. Non riusciamo a trovare una sola ragione, al di là dell'obbligo costituzionale della terza lettura, perché il Senato sia stati tenuto in ostaggio e messo nelle condizioni, durante l'intera sessione di bilancio, di rinunciare alle sue prerogative di indirizzo e di controllo. Se dobbiamo dirci la verità fino in fondo: se si è trattato di un esercizio muscolare, di forza, tutto interno alla maggioranza, e tra Governo e maggioranza; se non c'era nulla da cambiare in questa finanziaria, allora, a voler essere benevoli, oggi il Senato è stato chiamato semplicemente a farsi gli auguri. E anche noi dell'Italia dei Valori, una volta tanto, vogliamo adeguarci. Trasmettiamo gli auguri al Governo Berlusconi da parte delle famiglie italiane, che nulla o poco più di nulla hanno trovato in questa finanziaria. Auguri da parte di 2.600.000 famiglie che, secondo la cinica freddezza delle statistiche, si trovano in questo momento in condizioni di povertà relativa, perché il Governo affronta la crisi con una rete di protezione contro la povertà tra le più fragili nell'ambito dei Paesi d'Europa. Auguri da tutte le famiglie, perché c'è un dato più ampio e per questo meno visibile, che nasconde un livello di disuguaglianza sociale che descrive quanto sia difficile la condizione delle famiglie numerose, delle coppie con due o più figli, delle famiglie monogenitoriali, di quanto sia sempre più in salita in Italia creare una famiglia, diventare genitori, essere un giovane capofamiglia, in un Paese che negli ultimi anni ha scaricato sulle nuove generazioni i propri problemi economici e sociali. Tanti auguri al Governo Berlusconi da parte dei lavoratori che hanno perso o stanno perdendo i posti di lavoro e in questa finanziaria non hanno trovato nulla, o poco più di nulla, in termini di misure di sostegno economico e di politica industriale. Non è bastato l'allarme sociale dei lavoratori del gruppo Merloni (un gruppo di 3.000 dipendenti), una delle più gravi crisi industriali del Paese; non è bastato il previsto stop produttivo a Termini Imerese, la mobilitazione a Pomigliano d'Arco, con gli operai saliti sul tetto, e poi i dipendenti della Fincantieri di Sestri Ponente a Genova, di Muggiano a La Spezia e di Ancona, che da giorni dormono in cantiere. Non è bastata la grave situazione provocata dal blocco della produzione chimica degli impianti italiani a Porto Torres e a Marghera o i lavoratori in lotta da oltre un mese contro la chiusura dello stabilimento Yamaha di Lesmo (Monza). Tanti auguri da oltre un milione e mezzo di lavoratori atipici, ai quali è stato detto che in fondo sono fortunati perché i nostri sono i migliori ammortizzatori sociali e che allo stato delle cose con questa finanziaria possono contare nel migliore dei casi, se posseggono il terno al lotto dei requisiti richiesti, su una misura *una tantum* di 700 euro: una misura che ha visto fino a questo momento 15.000 domande all'INPS, di cui solo 1.500 accolte. Tanti auguri al Governo Berlusconi dal popolo delle partite IVA, dalle piccole e medie imprese, da un debole terziario falcidiato che da questa finanziaria, oltre ai miseri 200 milioni di euro per il credito d'imposta per l'innovazione, hanno visto nulla o poco più di nulla. Attenuare le tasse delle imprese sul lavoro, ridurre la burocrazia, sviluppare le infrastrutture materiali e immateriali non sono gentili concessioni, ma il meno che si possa pretendere da un sistema Paese degno di questo nome. Tanti auguri dai sindaci d'Italia, che pochi giorni fa hanno rotto il tavolo delle trattative con il Governo perché ancora una volta le promesse fatte sono state completamente disattese. Con le misure previste da questa finanziaria, dal mancato alleggerimento del Patto di stabilità all'ICI che viene restituita e neanche tutta, facendola passare come una misura eccezionale e non come quanto dovuto, i sindaci sanno che dovranno operare in condizioni ancora più difficili. Tanti auguri dalle donne e dagli uomini del Sud, che si sono illusi dell'annuncio fatto oltre tre mesi fa di un piano Berlusconi per varare una politica per il Mezzogiorno più complessiva e organica, per dare risorse nuove, attivare provvedimenti urgenti, sbloccare le risorse dei fondi FAS, e e invece alla fine hanno visto trasformare queste loro attese in una nuova banca per gli affari dei banchieri e una ricapitalizzazione della società Stretto di Messina spa tutta con denaro pubblico. Tanti auguri al Governo Berlusconi dai terremotati della Provincia dell'Aquila che ripagheranno tra breve le tasse per intero e, diversamente da chi le ha ripagate dopo dieci anni e solo al 40 per cento, si pagheranno così da soli la ricostruzione, anche perché gli appalti delle casette provvisorie sono costati, collega Lusi, 2.700 euro al metro quadro (rispetto alle previsioni di partenza di 1.200 euro) e qualcuno alla fine deve pur pagare. Tanti auguri al Governo Berlusconi dagli evasori, gli elusori, i falsificatori di bilancio, gli imbroglioni, i delinquenti che con lo scudo fiscale hanno fatto bingo, pagando solo il 5 per cento di quanto dovuto, sulla pelle e le tasche dei cittadini onesti che assolvono al loro dovere civico sino all'ultimo centesimo del loro sudato lavoro! *(Applausi dal al quarto Governo Berlusconi, perché dopo il quarto non vi sarà il quinto, in quanto gli italiani hanno già dato

Signor Presidente, colleghi, sono perfettamente consapevole che quello di oggi è un passaggio puramente rituale, perché in tempi - forse ormai residuali - di bicameralismo perfetto immaginare modifiche a questa legge finanziaria, per restituirla alla Camera nel periodo festivo, sarebbe davvero folle. Ma ciò non

In quella assise, addirittura, questo provvedimento è stato assistito dal voto di fiducia richiesto dal Governo; malgrado questo ulteriore elemento politicamente rilevante,

sia nella fase di predisposizione del testo (prima nell'ambito del Ministero dell'economia e poi nella sede collegiale del Consiglio dei ministri), sia durante il percorso parlamentare. È una legge blindata, alla quale la nostra partecipazione è stata denegata.

della maggioranza e che tuttavia viene costantemente espunto da essa. Un giorno, dovranno essere perfettamente ricostruite le ragioni che hanno determinato la scelta unilaterale del Governo e della coalizione

riconoscendo le condizioni di torto e il danno oggettivo sofferti dal Mezzogiorno in questo lungo processo di unificazione nazionale, che non si è certamente compiuto.

alla durezza dei conti e delle responsabilità di via XX Settembre, compie le scelte che attengono alla politica economica del Paese. In queste scelte, al di là di qualche annuncio

Abbiamo quindi ascoltato di un piano straordinario per il Mezzogiorno, annunci straordinari sul far dell'estate che invece, nella dura attività parlamentare autunnale ed invernale, vengono abbandonati,

Sa, signor vice ministro Vegas, a cosa somiglia la Banca per il Sud? A quegli specchietti che i *Conquistadores* offrivano ai poveri indigeni in cambio del loro tesoro. Il loro tesoro in quel caso era l'oro; il nostro è il consenso. Ci viene offerto uno specchietto per le allodole, anche se nessuno sa bene di cosa si tratti, ma sostanzialmente di questo dovremo accontentarci. Cos'è

Mancando dunque ogni altro preciso segnale in termini di scelte di Governo a favore del Mezzogiorno ed essendo mancata la possibilità di introdurre, anche per ragioni puramente estetiche, una qualsiasi nostra

È per queste ragioni che sinteticamente (senza voler tediare ancora l'Aula, visto che tutti abbiamo urgenze di tipo logistico), in piena coerenza con quanto già determinato dai miei colleghi della Camera, annuncio che i senatori del Gruppo Misto-Movimento per le Autonomie

ricordarne solo alcune, a memoria: pensiamo, ad esempio, ai confidi, al rifinanziamento importante dei contratti di produttività, agli incentivi per l'assunzione di ultracinquantenni e di lavoratori in cassa integrazione, al Patto per la salute; alla proroga per tutto il 2010 della cassa integrazione, un intervento assolutamente fondamentale, che da tanti era messo in dubbio.

Altri dati positivi li ricaviamo anche dall'approccio generale, e io devo, a questo punto, apprezzare sinceramente l'approccio dell'opposizione che nei suoi emendamenti ha trovato sempre delle forme di copertura

ci sembra il minimo. La seconda sfida, la più importante, è quella delle riforme. Ne stanno parlando tutti, ma non solo perché a Natale siamo tutti più buoni. La consapevolezza che le riforme sono ineludibili ormai dovrebbe avere colto chiunque.

in forma federale, affinché davvero noi possiamo avere uno Stato snello ed efficiente. È quello che possiamo permetterci: uno Stato al servizio dei cittadini e non cittadini al servizio dello Stato. *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa legge finanziaria, l'ultima dopo 31 anni, segna la conclusione di un ciclo economico e forse è destinata ad accelerare il mutamento degli scenari politici. La ripresa dell'economia mondiale è iniziata ma, per risalire la china e tornare ai livelli di prodotto, reddito e occupazione pre-crisi, occorreranno diversi anni (per l'Italia almeno quattro, secondo le più ottimistiche previsioni del Governo). Il contributo alla ripresa della nostra economia derivante dal complesso delle politiche attuate dal vostro Governo sarà, se le previsioni fragili saranno rispettate, solo dello 0,44 per cento: non lo diciamo noi, ma il vostro Documento di programmazione economico-finanziaria. Abbiamo ascoltato nell'anno e mezzo della crisi molti argomenti a sostegno della politica rinunciataria del Governo; tra i tanti con i quali il Ministro dell'economia ha supportato

per conseguire tale finalità, arginare il cosiddetto assalto alla diligenza in sede parlamentare. Mi chiedo e vi chiedo, signori della maggioranza: si può ragionevolmente ritenere che questi, pur minimali, obiettivi si siano realizzati? Non potete sostenerlo, perché non è vero. E non potete sostenerlo perché noi registriamo il più grave peggioramento dei conti pubblici degli ultimi 18 anni almeno: certo, per effetto della crisi, ma anche in conseguenza della politica del Governo.

Sempre la dura realtà ci dice che l'avanzo primario, il vero indice di virtuosità della politica di bilancio, precipita dal 2,4 per cento del PIL allo 0,4: un livello che non si registrava dal 1991. La spesa corrente primaria è salita in un anno del 3 per cento sul PIL, e non certo per effetto di manovre in deficit, che non sono state attuate (neanche per gli ammortizzatori sociali che sono stati attinti, com'è noto, da altri capitoli di bilancio), ma prevalentemente in virtù Qual è la concausa di questo peggioramento dei conti? Proprio quell'assalto alla diligenza che si voleva a tutti i costi evitare, non tanto in Parlamento, dove si è rifiutato qualunque confronto, ma all'interno stesso del Governo. In questi 20 mesi, i provvedimenti finanziari approvati, dal decreto ICI a questa finanziaria, sono stati nove. Sapete quanti sono i commi che compongono questi nove provvedimenti? Sono 2.520. Vi fornisco, se volete, le tabelle precise, redatte dai nostri preziosi collaboratori. Sapete quanti sono stati i commi delle leggi finanziarie del Governo Prodi? Lo stesso numero delle norme da voi approvate: Dunque, non è vero ciò che andate ripetendo da 18 mesi: mai più i film dell'orrore, roba da non proiettare più, dichiarava lo scorso anno il ministro Tremonti a proposito delle vecchie finanziarie (anche delle sue). Sennonché, il film è stato ugualmente proiettato, eccome, in nove puntate, ma la trama, gli attori, la scenografia sono stati scelti non sotto gli occhi degli italiani, qui in Parlamento, nel fuoco del confronto democratico, ma nelle stanze dei Ministeri, di pochi Ministeri.

con la non banale differenza che noi avevamo un senatore in più, e non sempre; voi 50 senatori e 100 deputati in più. Dentro questo scadimento del rapporto Governo-Parlamento, qui al Senato, signor Presidente, di quei nove provvedimenti (sei decreti, due finanziarie e un collegato), ben cinque sono usciti senza modifiche, due con limitatissime variazioni. Con questa finanziaria si è prodotto il massimo della forzatura regolamentare; entra dal Governo con 30 commi, esce con 68 da quest'Aula del Parlamento; alla Camera si votano in Commissione 200 emendamenti in 10 minuti; tutto si conclude con un maxiemendamento non del Governo, sul quale porre la questione di fiducia, come pure prevede la Costituzione, ma del relatore: una innovazione fantasiosa, con la quale la finanziaria è stata riscritta *ex novo*, balzando quindi a 266 commi, e senza discussione alcuna. E al Senato, naturalmente, come abbiamo visto, una nuova blindatura. Questi sono i risultati di 20 mesi di manovrette adottate senza una strategia e sotto il segno della prudenza. Ma che politica economica è quella messa in atto dal Governo? A quale modello e principi si ispira? In Europa, oltre al sostegno alle fasce deboli della popolazione, sono state mobilitate ingenti risorse per gli investimenti pubblici e per i settori strategici dell'economia. Da noi, si è oscillato tra una nuova teorizzazione interventista dello Stato al quasi niente. E invece avevamo bisogno di una manovra robusta

e riformando il sistema degli ammortizzatori sociali; di sostenere l'occupazione (oltre 500.000 posti di lavoro sono stati persi questo anno) con il credito di imposta automatico, gli investimenti in ricerca e e innovazione e riducendo selettivamente l'IRAP, allentando il Patto di stabilità interno. Si trattava di sostenere gli investimenti pubblici e privati orientandoli verso l'economia verde di cui abbiamo urgente bisogno, la sicurezza degli edifici, del territorio, delle persone. E invece siamo passati dalla *social card* e dal *bonus* famiglie (che i cittadini italiani stanno dimenticando molto in fretta) ad una manovra, quella che oggi voterete, fatta di molte cose inutili e di altre misure obbligatorie, e coperta in gran parte dalle entrate dello scudo fiscale (proventi di attività illecite) e dallo sconsiderato utilizzo del TFR dei lavoratori (fu un errore che commise anche il Governo Prodi ma almeno in quel caso furono finanziati solo investimenti; oggi utilizzate il denaro dei lavoratori per finanziare la spesa corrente). Una politica caratterizzata da una costante, quella dello sperpero delle sole risorse stanziate nel 2007 per il Mezzogiorno e le altre aree in difficoltà, il FAS nazionale, 27 miliardi in 7 anni che dovevano sostenere la crescita del nostro Paese e che invece stanno percorrendo mille rivoli. Ma voi, signori del Governo e della maggioranza, state perdendo la sfida sul vostro terreno dì gioco. Volevate meno pressione fiscale e abbiamo più pressione fiscale (arrivando al livello record del 43,4 per cento). Volevate meno spesa corrente e più investimenti e abbiamo l'esatto contrario (ieri il senatore Giaretta ed oggi il senatore Marco Filippi hanno fornito dati inequivoci sul crollo degli investimenti pubblici); volevate più risorse e mezzi per la sicurezza e invece i nostri carabinieri, poliziotti, vigili del fuoco stentano ad ottenere le risorse per i mezzi, il carburante e gli straordinari. Una crisi identitaria, come è stata definita dalla presidente Finocchiaro, in occasione della prima lettura di questa legge, che ha prodotto le prime vistose crepe nella maggioranza, qui in quest'Aula dove importanti emendamenti alla prima lettura non passarono solo per la disposizione regolamentare sul computo dei voti di astensione. C'è un'Italia che soffre, che non ha i mezzi per sopravvivere, ci sono i giovani ai quali lasciamo più debito e meno futuro. A loro questa finanziaria non parla. Ma c'è anche un'Italia che che reagisce, che studia, che lavora per la propria famiglia e per la collettività, che fa impresa innovativa e competitiva. Quell'Italia migliore che non si riconosce più nelle vostre politiche e nelle vostre decisioni. Quell'Italia alla quale abbiamo provato a rivolgerci nel formulare le molte proposte che vi abbiamo sottoposto, per le quali ci siamo battuti e che avete sistematicamente respinto, anche qui oggi in quest'Aula. Infine, signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo vicini a Natale. Consentitemi di chiudere con un richiamo al terremoto abruzzese. Siamo passati da un efficace intervento nella fase di emergenza, che abbiamo apprezzato, per il quale per il quale dobbiamo ringraziare Protezione civile, volontari e popolazione locale, ad un massiccio uso mediatico di quella tragedia per celebrare supposti record mondiali dell'azione di governo. Signor vice ministro Vegas, per favore, non dite più che non è mai stato fatto di meglio in casi come questo, perché non è così. Ad oggi, dopo quasi nove mesi, 16.000 cittadini sono ancora negli alberghi, e lì passeranno il Natale. La ricostruzione vera non è iniziata e con questo provvedimento state predisponendo la più odiosa tra le misure, quella di imporre la ripresa del pagamento delle imposte e contributi a partire da gennaio, una misura insostenibile per chi è ancora senza casa, senza lavoro e senza azienda, tanto che il Governo si sta affannando, in queste ore, a ricercare una soluzione con il decreto milleproroghe. Può darsi che una misura parziale sarà individuata, ma per favore non utilizzate più il terremoto per esaltare i successi del Governo. Non fate più promesse che non potete mantenere: mantenere: né ai terremotati, né ai destinatari della *social card*. Cambiate politica, il Paese ne ha un bisogno urgente. Per queste ragioni, signor Presidente, e per quelle che abbiamo ampiamente illustrato nel corso della sessione di bilancio, voteremo convintamente contro questa manovra.

alla sessione di bilancio possa condurre a migliori risultati sia l'azione del Governo sia l'azione del Parlamento. Voglio ora soffermarmi

Taluni, invece, specie dopo il ritorno della legge dalla Camera, si sono soffermati sulla quantità di misure che il Governo ha adottato, parlando di eccesso di spesa. Secondo me la questione è totalmente mal posta. La verità è una,

ai fini del bilancio dello Stato - la manovra è espansiva, e lo è esattamente per le seguenti

2012. In questo momento, quindi, come avevamo già detto alla fine della prima lettura, questo provvedimento completa il disegno del Governo attraverso una manovra che, nei limiti consentiti dalla nostra situazione finanziaria, rende possibile tentare due operazioni importanti: in primo luogo, alleviare i morsi della crisi sui ceti più deboli e, in secondo luogo, tentare di attendere la ripresa al varco, consentendo di cogliere le opportunità che da essa saranno offerte. Questo è il dato che emerge dalla manovra. Per la verità, in questa manovra, esiste un problema, che però non attiene all'attuale situazione ma a quella che affronteremo. Infatti, se è vero che la manovra è espansiva ai fini del saldo netto, è altrettanto vero che essa è neutrale ai fini dell'indebitamento netto. Questo è un problema che pone delle domande a proposito della nuova sessione di bilancio e delle nuove sfide che dobbiamo affrontare.

a seguito della crisi, sia cresciuta in misura notevolmente inferiore a quella di tutti gli altri Paesi occidentali, anche di grandi *competitor* come la Germania o la Spagna.

All'interno di questo ragionamento era stato detto che, siccome le spese erano possibili soltanto nell'ambito e nella misura delle risorse provenienti dallo scudo fiscale, esse,

tra il Governo e il Parlamento, perché alla fine gli elementi di ragionevolezza emersi nel corso del dibattito sia in Commissione che in Aula avrebbero potuto sortire effetti migliori. Faccio appello perché si comprenda fino in fondo che l'attività parlamentare va affrontata con grande serenità e che tale questione mediatica dell'assalto alla diligenza è qualcosa che non c'è più nel nostro rapporto. È infatti da tempo che l'articolo 1 della legge finanziaria si approva prima di tutti gli altri e che quindi all'interno di quei saldi determinati si compie l'intera manovra. Questo è il dato di fondo di cui dobbiamo si deve migliorare il rapporto. La nuova sessione di bilancio lo migliorerà, ma oggi, in questo quadro, la finanziaria completa una manovra che ha dei limiti, ma anche dei pregi di fondo: il nostro PIL scende meno che in altri Paesi, la nostra inflazione è sotto controllo,

Non solo, abbiamo affrontato anche i problemi minori. Non sono d'accordo che per l'ordine e la sicurezza pubblica non è stato fatto niente. È esattamente il contrario: sono state appostate significative risorse per le nostre forze dell'ordine,

ci si pone ancora il problema del rilancio delle iniziative infrastrutturali come una delle opzioni per poter sostenere la ripresa. Questo è il dato di fondo entro il quale la manovra finanziaria si inscrive. Certo, ci sono poi piccoli interventi, che io non che io non disprezzo, perché anch'essi sono di una certa efficacia e, quando questi riverberano i loro effetti positivi su comunità di lavoro anche piccole,

a favore della legge finanziaria, auspicando un migliore rapporto tra Governo e Parlamento, certi di aver fatto il meglio possibile in queste condizioni, determinati a condurre l'azione di governo in materia economica e di finanza pubblica nel 2010 tenendo fermo il discorso del non aumento del debito pubblico, con un tentativo di risanamento del rapporto tradeficit e prodotto interno lordo e con la chiara coscienza che non sarà più possibile agire